Presidente, credo che dovremmo riflettere sul processo verbale che si sta per approvare perché non è stato menzionato in modo corretto o comunque in modo chiaro quanto è accaduto ieri sera in conclusione di seduta. ieri sera in conclusione di seduta. Ieri sera abbiamo evidenziato un problema di straordinaria importanza.

dovrà, infatti, verificare esattamente cosa è stato scritto e se è stato correttamente riportato un dibattito, sia pure a fine

Cisiamo trovati di fronte al fatto completamente nuovo di un emendamento, proposto dalla Commissione,

parlare delle modalità di espressione del voto in quest'Aula. Anche ieri sono stati commessi diversi abusi, che hanno dato luogo a vivacissime contestazioni e che solo per miracolo non sono diventate vere e proprie gazzarre, come avvenuto in altre votazioni in questa Aula. Ora, io e molti altri colleghi riteniamo che nei costi della politica ci sia anche l'erosione della fiducia dei cittadini quando essi si accorgono che le regole non sono seguite, che vi sono abusi nell'espressione del voto: sanno che ogni voto dato fuori delle regole erode questa fiducia ed ha un elevatissimo costo politico. Il costo della politica risiede anche in questo. Ritengo che anche l'assegnazione di un posto fisso non risolva il problema dell'abuso. L'unico modo di risolvere per sempre, alla radice, l'abuso nell'espressione del voto è adottare un sistema di voto digitale. Questo sistema non consente la duplicazione, consente l'espressione del voto da qualsiasi postazione, è un sistema sicuro ed economico.

in ambedue gli schieramenti. Nell'opposizione hanno sottoscritto la lettera persone di rilievo, come lei, presidente Calderoli, o come il presidente Matteoli. Se ci sono più firme dai settori della maggioranza che da quelli dell'opposizione dipende solo dalla mia maggiore dimestichezza con questo lato dell'Aula e dalla minore dimestichezza che ho con con l'altro lato; sono però sicuro che se mi dessi da fare per un'altra mezza giornata queste 160 firme diventerebbero 300. Non ho ancora ricevuto risposta a questa lettera,

Signor Presidente, ieri sera, nella seconda parte del TG2 delle 20,30, è andato in onda un servizio sulla Rivoluzione d'ottobre. Affermo in modo determinato, forte e chiaro che questo è stato un servizio vergognoso. È stato esplicitamente detto, signor Presidente, che la Rivoluzione d'ottobre è stata solamente un sanguinoso colpo di Stato, che ha messo fine alla vera rivoluzione, quella menscevica, che ha prodotto solo un nuovo zarismo; che ha gettato la Russia nel sangue e nella violenza; che ha esportato con la forza l'orrore nel mondo *(Proteste dai banchi dell'opposizione)*; che la Rivoluzione d'ottobre ha favorito il sorgere del fascismo in Italia; che lo stesso nazismo sarebbe nato per combattere il mostro del comunismo;

E per dare forza a tale affermazione*,* il servizio si è chiuso con le immagini di manifestazioni operaie italiane degli anni Sessanta con le bandiere rosse. ironici dai Gruppi LNP, FI, UDC e AN)*, come si alzavano in piedi i contadini di Di Vittorio di fronte ai padroni delle terre. Mi sono alzato in piedi, senza togliere il cappello, per dire a tutti che questo servizio televisivo è stato contro la democrazia, contro la storia e contro la civiltà.

Ha dimostrato che lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sulla donna non è un destino ineluttabile; che i padroni, come l'aristocrazia francese, non sono figli di Dio.

e le grandi lotte operaie e contadine di questo Paese furono possibili anche grazie all'ideale acceso dalla Rivoluzione d'ottobre. Il comunismo, si è detto, sarebbe uguale al nazifascismo: si vergognino!

e come i nazisti di un tempo hanno in odio i diversi, i rom, gli immigrati, i comunisti. Noi, i comunisti e la sinistra, come sempre, per nostra natura, per nostro ideale, siamo dalla parte della pace e dei lavoratori *(Vivi, ironici*

Purtroppo gli studenti delle scuole vengono generalmente indottrinati con quella grottesca visione della Rivoluzione d'ottobre e di altri avvenimenti del genere che invece ci ha riferito il senatore Giannini. Per ricordare alcuni dettagli, nei soli cinque mesi seguiti alla Rivoluzione d'ottobre ci sono state più uccisioni e più condanne a morte, senza contare quelle extragiudiziali, che negli ultimi novanta anni del regime zarista. La Rivoluzione d'ottobre non è stata, come generalmente viene detto ai nostri studenti, una rivoluzione contro lo Zar, ma una rivoluzione contro la nascente repubblica democratica che si stava instaurando in Russia. *(Applausi dai Gruppi che causa indignazione le poche volte in cui lo si sente. Dovremmo, questo filmato, ma soprattutto questa verità, farla sentire anche nelle scuole, perché i nostri studenti sono sottoposti ad un indottrinamento tale che forse alcuni di loro si sono sdegnati, come si è sdegnato, completamente a torto, il senatore Giannini.

dalla RAI, perché gli italiani devono sapere chi i senatori a vita, i cosiddetti moderati alla Follini e quant'altri

perché il giudizio sulla Rivoluzione d'ottobre è ancora una discriminante fondamentale nella politica del nostro tempo. È difficile negare che essa sia stata una rivoluzione contro un Governo democraticamente eletto,

ma un'opinione largamente diffusa nella storiografia e che porta la firma di una grande vittima e testimone del dramma del comunismo, cioè Alexander Solgenitsin. Ricordo

generato prima il comunismo e poi il nazifascismo, perché come la storiografia moderna più accreditata ha riconosciuto (voglio qui ricordare gli studi di Renzo De Felice in Italia, ai quali io ho preso parte in maniera modesta ma, a quel tempo, non disprezzabile), il fascismo nasce come risposta al comunismo. Non vi è una giustificazione del comunismo come lotta anti fascista, ma è il contrario! Il nazionalsocialismo è anch'esso una risposta al comunismo, che tenta di superarlo in orrore (e forse vi riesce), ma partendo dalla medesima impostazione fondamentale. Davanti a questo orrore, si erge la resistenza della coscienza dell'Europa. Non si può parlare di comunismo senza ricordare Lech Walesa, senza ricordare *Solidarność*, senza ricordare Giovanni Paolo II, perché quell'orizzonte di violenza e distruzione

Sapete cosa vuol dire non poter parlare liberamente neanche all'interno della propria cerchia famigliare, per il sospetto che vi sia una spia? Sapete cosa vuol dire che l'amico, il compagno, il fratello possono essere trovati morti (perché i casi come quelli di don Popieluszkosono stati tanti)

Vogliamo parlare del comunismo? Vogliamo discutere dell'equivalenza morale di comunismo e nazionalsocialismo con la realtà dei fatti? Credo sarebbe opportuno, signor Presidente, che questo Senato dedicasse una volta una sessione di studio a riflettere sulle radici della politica contemporanea. La lotta per la libertà è indissolubilmente lotta contro il nazifascismo, lotta contro il comunismo e lotta contro il totalitarismo. Questa è la verità su cui si regge la democrazia occidentale e su cui si deve reggere anche la democrazia italiana.

hanno combattuto il nazifascismo alleandosi con Hitler per aggredire la Polonia con il patto Ribbentrop-Molotov, quindi per ben due anni il comunismo sovietico è stato alleato fedele dei nazisti. Così ha combattuto la Rivoluzione d'ottobre il nazionasocialismo e il fascismo! Non solo: poi ci furono i massacri come la fossa di Katyn dove furono uccisi e massacrati decine di migliaia di ufficiali dell'esercito polacco per decapitare la borghesia e il ceto medio polacco. Questa è stata la Rivoluzione d'ottobre in Polonia e non solo in Polonia. Ora, Presidente, voglio soffermarmi su quanto sta avvenendo a Napoli.

è ripreso nel quartiere di Pianura, in cui furono massacrati due studenti cinque anni fa, innocenti ed estranei alla guerre tra cosche criminali, criminali, il massacro in quanto la magistratura napoletana ha ritenuto di liberare tre esponenti di primo piano di uno dei *clan* più sanguinosi della Campania, il *clan* Lago. Questo avviene nel momento in cui la procura di Napoli ritiene di insabbiare una denuncia per estorsione avanzata dall'imprenditore Antonio Supino, quale da circa quattro anni è alle prese con il *clan* Lago che gli vuole impedire di aprire un parcheggio auto per 500 posti. Bene, questa denuncia è stata insabbiata e il consulente *antiracket* della Regione Campania, e poi del Comune di Napoli, a una richiesta di aiuto dell'imprenditore Supino ha risposto, nel momento in cui presentava le denunce contro i camorristi: che cosa poteva aspettarsi, che gli portassero i cannoni a casa? Questo è il clima di quella città. Le chiedo, signor Presidente (non so se sia qui presente il Ministro della giustizia), di avere una risposta informata a quanto sto dicendo oggi, cioè che nella procura di Napoli giacciono inevase denunce con nomi e cognomi contro gli estorsori di questo *clan* e nessuno fino ad ora ha mosso un dito. Non solo: l'imprenditore Supino, sottoposto a minacce, è stato colto da infarto cardiaco. Ora, se l'imprenditore Supino subirà la stessa sorte di questo lavoratore massacrato ieri a Pianura, si sappia in quest'Aula che la responsabilità è dei magistrati e della procura di Napoli che ha insabbiato la sua denuncia.

Rivoluzione d'ottobre, io non credo che una seduta possa esaurire un argomento del genere. Oggi noi abbiamo all'ordine del giorno un decreto che comunque reca misure importantissime, che piacciano o non piacciano, per il Paese. Questa è la strada migliore per non riuscire a votare le proposte dei senatori della Commissione e andare dritti alla fiducia. Io credo che sia interesse di tutti

Avevamo cercato di affrontare nuovamente un problema che nella passata legislatura e anche prima ha costituito motivo di dibattito e di confronto dialettico all'interno dei due rami del Parlamento, che è quello delle cooperative. I colleghi e il Presidente ricorderanno che, rispetto allo scenario mondiale delle società e quindi del rapporto che nasce tra due o più persone per mettere insieme beni, capitali o servizi al fine di conseguire un lucro, accertata la professionalità degli stessi e quindi la non occasionalità, la persecuzione del lucro registra una eccezione nel nostro ordinamento, perché quel lucro non è una conseguenza assoluta sicura e riconducibile a quello che avviene nelle altre parti del mondo, atteso che esiste una particolarità di impresa che è quella delle cooperative.

per esse deve essere applicato il medesimo sistema impositivo esistente per le imprese, per il capitale, direi per i padroni, a sentire l'illustre senatore Giannini, che nel suo intervento ha rilevato di non essere un uomo qualunque, ma di essere il comunista che esiste sempre nelle vostre file. Se vogliamo fare una cosa seria, bisogna allora dire "basta" a questa ipocrisia: le cooperative, quando vogliono scalare le banche, non sono più tali e, superata una certa soglia, benedetto Iddio, paghino le tasse! Questa è la nostra proposta, ma voi non avete il coraggio di accettarla, perché siete ancora vincolati da una retriva imposizione che è quella di una società statalista. *(Applausi

distribuzione del testo non è sufficiente se non abbiamo il tempo anche di esaminarlo. Se continuiamo i nostri lavori, non siamo capaci di fare due cose insieme: siamo modesti personaggi e possiamo fare una cosa alla volta.

il relatore, in rapporto con il Governo e con la maggioranza, sta cercando di vedere se c'è una soluzione da presentare, diversa dai testi al nostro esame, che possa raccogliere le diverse esigenze che si accumulano che si accumulano in maniera contraddittoria attorno a questo tema. È del tutto evidente che c'è nella maggioranza un problema, non è che bisogna essere particolarmente acuti per cogliere tale aspetto.

può accadere di avere bisogno di mezz'ora di tempo per definire una scelta politica. maggioranza, approvando la richiesta del relatore di accantonare gli emendamenti relativi alla vicenda «Ponte sullo Stretto». Noi avevamo manifestato la nostra contrarietà chiedendo che l'Aula si pronunziasse sulle proposte emendative. L'Aula, sovrana, ha deciso di accantonarle. accantonarle. La decisione della Presidenza, della quale abbiamo preso atto, era quella di tornare immediatamente al voto su questi argomenti alla ripresa dei lavori, cosa che, puntualmente, la Presidenza sta realizzando. Adesso la maggioranza dichiara di non avere ancora, nonostante la serata, la notte e la mattina, risolto questo problema. Ebbene, noi siamo all'opposizione abbiamo assunto una posizione responsabile in quest'Aula sulle votazioni relative a questo decreto-legge, ma non siamo certo un'opposizione stampella di una maggioranza che non c'è più. Allora, insistiamo, visto che c'è stato tanto tempo perché il Governo e la maggioranza risolvessero al proprio interno la questione,

valutare la posizione da assumere. Se però questo emendamento non c'è, non si possono paralizzare i lavori dell'Aula in attesa che la maggioranza risolva i suoi storici e strutturali problemi. Signor Presidente, manifesto la piena contrarietà alla richiesta di sospensiva anche perché questo tema - ripeto - è stato già affrontato ieri, anche con una sospensione dei lavori. Credo sia giunto il momento, davanti agli occhi di tutti, che il Governo e la maggioranza ci dicano cosa intendano fare di una società che ha stipulato un contratto di appalto con un imprenditore, sottoposto alle regole del diritto civile, se questa società committente intende liquidarla per decreto, quindi per atto di imperio, o se intende rispettare il nostro codice civile e le aspettative di operatori internazionali che hanno investito e stipulato un contratto correttamente

C'è stato il tempo per ragionare, per trovare soluzioni. A mia conoscenza e a conoscenza dell'Italia dei Valori, soluzioni, in questo momento, non ve ne sono. Pertanto, credo che un ulteriore rinvio, non propedeutico e non costruito, non gioverebbe all'interesse del Paese.

La seduta è ripresa. Invito i colleghi a prendere posto.

poi è diventato professore di storia contemporanea: è stato uno dei grandi storici dell'età contemporanea che il nostro Paese abbia avuto, forse forse il maggior storico del movimento cattolico in Italia. Ma è stato anche un protagonista della vicenda politica italiana: è stato senatore, animatore della sfortunata Commissione bicamerale Bozzi sulle riforme costituzionali

il professor Scoppola sia mancato due giorni prima dell'Assemblea costituente del Partito Democratico.

Presidente, mi scusi l'insistenza, però, visto che in alcuni casi la storia viene strumentalizzata, ce ne sono altri nei quali essa può servire anche per scrivere una pagina di civiltà. civiltà. Come schieramento vogliamo unirci al cordoglio che ha espresso il senatore Tonini per la scomparsa del senatore Scoppola.

fondamentali della nostra storia comune, lo ha fatto anche esponendo tesi - che molto spesso non sono state gradite e sono state contrastate da storici che avevano idee diverse diverse - con una civiltà e un rispetto che credo facciano parte non solamente del nostro patrimonio culturale ma anche del nostro patrimonio istituzionale. Dirlo oggi al momento della sua scomparsa e dopo che così male avevamo aperto i lavori questa mattina credo sia un modo per recuperare la sua memoria, che fa anche onore alla nostra istituzione.

ho fatto parte nel corso degli anni Settanta di quel tentativo di rinnovamento della Democrazia Cristiana che ebbe luogo attraverso i cosiddetti esterni della Democrazia Cristiana ed ebbi l'onore di essere votato da Scoppola come rappresentante degli esterni nel rinnovamento della Democrazia Cristiana.

Qui termina il mio ricordo personale, che si intreccia con quello politico. Pietro Scoppola è stato, lo ricordiamo, un grande interprete della grande stagione dei cattolici al Governo del Paese. Da questo punto di vista le opinioni, che possiamo non aver sempre condiviso, hanno rappresentato e rappresentano uno straordinario contributo per la conoscenza della storia del nostro Paese. *(Applausi)*. Colleghi, non volevo assolutamente limitare il cordoglio, credo sia un argomento estremamente importante. Purtroppo, questo Parlamento, non so se a ragione o a torto, tratta di tutto meno che di quello che dovrebbe trattare, Grazie,

un segmento importante della Repubblica italiana e della nostra Costituzione, un grande storico, un grande studioso, un cattolico democratico, che personalmente è stato anche parte della mia modesta formazione giovanile. Una persona che ha ritenuto che i grandi partiti, le grandi organizzazioni democratiche, la Democrazia Cristiana come il Partito Comunista, siano stati veicolo di democrazia, siano stati

del professor Scoppola dà l'occasione di indagare e di pensare seriamente a cosa è stata una stagione in cui i cattolici organizzati, i cattolici democratici e i comunisti organizzati sono stati l'architrave della costruzione della Repubblica antifascista, della Repubblica che ha saputo uscire dal nazismo, dal fascismo e dalla guerra. Per questo vogliamo ricordare una grande figura, non

(con lui Bobbio e molti altri) che hanno partecipato su più versanti, magari dialettici tra loro, ma hanno contribuito tutti alla costruzione di quell'*ethos*, di quella cultura di massa, di cui il nostro Paese oggi può vantare la priorità anche in Europa. Quindi, ringraziamo Scoppola, ringraziamo il cattolicesimo democratico, ringraziamo una cultura che è parte integrante della storia e dell'attualità repubblicana e antifascista del nostro Paese. SALVI *(SDSE)*. A nome mio personale e del Gruppo della Sinistra Democratica mi associo al lutto della famiglia e del Paese per la scomparsa di Pietro Scoppola, grande e acutissimo storico della Prima Repubblica, personaggio di primo piano del cattolicesimo democratico e figura di specchiata etica pubblica e personale. Lo ricordiamo con commozione in questo momento. anche a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale esprimo il cordoglio per la morte Di Pietro Scoppola, ricordandone le qualità umane e culturali. È morto un grande storico. Pur non condividendo la lettura del cattolicesimo di Pietro Scoppola, certamente non possiamo non rimpiangere questo personaggio che è stato soprattutto un grande galantuomo e un grande uomo di cultura. desidero esprimere l'emozione del Gruppo che si intitola alla Democrazia Cristiana per la scomparsa di un personaggio che nella cronaca di oggi si collega all'esperienza del nascente Partito Democratico ma che nella storia dalla cultura politica italiana entra, e resta, per il volume che è negli scaffali di tutti gli appartenenti alla mia generazione:

che porta la sinistra italiana oggi e qui a dire le cose belle, che io condivido, che abbiamo ascoltato dal collega Russo Spena. l'emozione per la scomparsa di Scoppola, per onestà intellettuale, non deve distrarci dalla constatazione che non sempre la sinistra italiana ha detto di De Gasperi le cose che dice oggi. Forse la grandezza intellettuale e politica di Pietro Scoppola è stata proprio la capacità di documentare la straordinaria figura di Alcide De Gasperi e l'azione della Democrazia Cristiana nel dopoguerra con una tale dovizia di particolari e di argomenti da convincere la sinistra italiana di tradizione comunista a dissociarsi dai luoghi comuni con cui aveva alimentato decenni di comizi e a convergere su un giudizio storico che, seppur con qualche tratto di opportunismo, completa la collocazione di De Gasperi nel *pantheon* di coloro che meritano a pieno titolo l'appellativo, spesso purtroppo abusato, di statisti. Con questo pensiero, che piacerebbe al professor Scoppola perché forse un po' rude ma vicino alla sua abitudine intellettuale ad evitare la retorica, mi unisco al generale cordoglio per la sua scomparsa, che priva il Paese di una delle sue coscienze più alte.

e lui era uno straordinario storico laico, profondamente laico, e rispettoso delle idee. Mi ha insegnato moltissimo; abbiamo avuto tantissime discussioni, ma non ho mai sentito nessuna diversità fra me, comunista ed atea, e lui, cattolico ma profondamente laico, dotato di un senso dello Stato, delle istituzioni e di una lettura della storia che volava così alto che sentirlo

notizia della scomparsa di Pietro Scoppola con un senso di angosciosa amarezza e sorpresa, date le occasioni - anche recentissime - di incontro e di collaborazione avute insieme.

perché egli è stato un grande intellettuale della cultura politica dei cattolici nel nostro Paese. I suoi studi sul pensiero cattolico, sulla storia dei cattolici politicamente impegnati e sulla interpretazione data dalla cultura cattolica alla storia italiana resteranno fondamentali per i cattolici; ma anche per i laici, come ha detto prima di me la senatrice Palermi. Egli era una personalità

dalla sua frequentazione, dalla grande apertura mentale che lo distingueva. Ad accomunarci abbiamo abbiamo avuto l'interesse per il passato e per il futuro. L'interesse per il passato, perché egli è stato, come già altri hanno detto, un grande storico della Repubblica.

è stata scritta da Pietro Scoppola. Dunque credo che questo sarà il primo dei suoi scritti postumi ad essere pubblicato e una delle sue ultime opere di interpretazione storiografica. Oltre ad essere stato un grande storico della prima Repubblica, se così si vuol chiamare la Repubblica dei partiti usciti dalla liberazione, Pietro Scoppola è stato anche un grande

la carta dei principi del partito di "democrazia è libertà", la Margherita. Scoppola è stato poi sempre un referente culturale di primo piano nel processo di costruzione del nuovo partito: il partito democratico che compie ora il suo esordio, e di certo avrebbe avuto grande vantaggio dalla sua opera, dal suo pensiero, dal suo insegnamento, dalla sua testimonianza. Lo ricordo con sincero

Pietro Scoppola fu un senatore indipendente della Democrazia Cristiana in una particolare stagione, per la verità non felicissima, i cui esordi

Scoppola va ricordato come storico. Esordì con alcune partecipazioni agli eventi della storia italiana facendo cenno al passaggio al neoguelfismo, alla Democrazia Cristiana. L'ultimo dei suoi libri tratta la democrazia dei cristiani, con considerazioni che, per quanto mi riguarda e con l'affetto che mi maturava e che sottoponevo come giudizio nelle occasioni in cui c'era incontro, non sempre condividevo. Però mi inchino reverente alla sua memoria come cattolico. Lo fa il Governo nella sua laicità, perché oggi è morto un grande storico, un uomo impegnato nella cultura italiana senza alcuna aggettivazione. Il Governo è solidale con la sua famiglia e con quanti gli sono accanto.

per una perdita che consideriamo del Paese. La consideriamo una perdita di tutti perché Pietro Scoppola è stato un intellettuale di tutti. È stato l'intellettuale che, ponendosi da un punto di vista cattolico, ha tuttavia suscitato un grande e continuo dibattito in ordine al processo di sviluppo della democrazia nel Paese; quindi, un cattolico che ha contribuito molto allo sviluppo di uno Stato democratico e liberale. Lo ricorderemo come un esempio di senso dello Stato, di di uomo di cultura alta che media continuamente fra i valori del cattolicesimo e del cristianesimo e i valori liberali della laicità dello Stato. Noi pensiamo che questo Paese, nella fase evolutiva della politica, abbia tratto molto dall'ingegno di Pietro Scoppola. Noi della Lega Nord, che conosciamo, e siamo abituati talvolta silenziosamente a custodire nel nostro animo e nelle nostre menti, il contributo di coloro che hanno partecipato seriamente

manifestare la volontà di non incorrere nella cosiddetta ghigliottina; credo che negli interventi che seguiranno sia interesse di tutti non arrivare a quella procedura che - ricordo - determinerebbe il voto senza interventi solo degli emendamenti approvati in Commissione. Credo che questo rappresenterebbe il massimo danno per l'Assemblea. Il presidente Morando Sì, signor Presidente. La Commissione si è riunita, su suo mandato. È stata messa in votazione la proposta del relatore

Presidente, dopo la comunicazione del presidente Morando, per venire incontro alle esigenze di brevità, ma anche perché ritengo che la situazione interna alla maggioranza consenta

relativo alla viabilità secondaria nelle Regioni Sicilia e Calabria, potrei ritirarlo e trasformarlo in un ordine del giorno, atteso che l'argomento sarà certamente ripreso nella prossima finanziaria. Si tratta - come ho detto nel mio intervento di ieri - di una prescrizione di legge allo stato non

Il punto di riferimento dell'Italia dei Valori in questa vicenda è e resta il provvedimento uscito dal Consiglio dei ministri, sul quale ci attestiamo e verso il quale manteniamo una posizione di fiducia. Ci sembra che non si sia svolto un buon lavoro e soprattutto che questo emendamento, purtroppo, esponga ad azioni di responsabilità civile verso il Paese - così come veniva in precedenza evidenziato

dei contratti. Chi sostiene che questo è un modo per buttare via risorse pubbliche mente. Conosciamo tutti le regole e i contratti; ho qui una lettera del presidente della società Ciucci, ora anche amministratore dell'ANAS, nella

in nome di questa importante affermazione dell'amministrazione delegato, abbiamo assunto questa decisione difficile. Naturalmente non credo che lasciare in un cassetto un contratto significhi ridurre in futuro il contenzioso. Ci siamo resi disponibili ad altre mediazioni, che però non hanno convinto altre parti della maggioranza; credo che questa sia una soluzione accettabile e giusta per dare una soluzione di prospettiva. di prospettiva. Abbiamo già destinato a Sicilia e Calabria 1 miliardo di euro per infrastrutture che servono e, con la parte dell'articolo 8 che abbiamo sostanzialmente già votato (perché gli emendamenti sono stati respinti), stanziamo

di mobilità dell'area dello Stretto. Per queste ragioni, chiedo ai colleghi di votare a favore dell'emendamento 8.701 della Commissione.

Il testo è stato adottato dalla Commissione dopo una discussione lunga e approfondita. Esso, ovviamente, non viene condiviso - dico ovviamente perché il senatore Formisano lo ha appena annunciato - da da una delle forze che compongono la maggioranza ed il Governo ne ha chiesto il ritiro, fermo restando l'impegno della Presidenza del Consiglio a formularne uno ulteriore.

la costituzione di un sistema di trasporto intermodale che garantisca il collegamento tra il Mezzogiorno, in particolare la Sicilia, e il resto d'Italia. È ovvio che questo testo nella sua vicenda parlamentare ha visto la disponibilità di tutta la maggioranza a trovare ulteriori soluzioni che potessero essere più soddisfacenti e consone alle aspettative dell'intera maggioranza. Così è stato con l'accantonamento del voto di ieri per consentire un ulteriore approfondimento e così è stato oggi, con la responsabile richiesta da parte della Presidenza del Consiglio di prendere ancora altro tempo. Credo che potremmo, però, convenire che di fronte ad una così inequivoca manifestazione di volontà da parte della Commissione bilancio e della maggioranza in quella sede, ferma restando la piena apertura e disponibilità ad una rivalutazione del testo e della sua costruzione, il voto del mio Gruppo non possa che essere favorevole.

non del tutto soddisfacente, ma che comunque raccoglie il consenso e gli spunti fondamentali sui quali il dibattito si èconcentrato.

La soluzione adottata dalla Commissione chiude definitivamente la questione del ponte sullo Stretto di Messina. La chiude e non determina, a differenza di quanto sostenuto, aggravi a carico del bilancio dello Stato che già non esistano in questo momento. Infatti, se così fosse, gli aggravi si sarebbero dovuti determinare già nell'ambito del giudizio che la Commissione ha espresso su questo emendamento,

ci sarà un voto che accoglierà compiutamente questo emendamento, potremo dire che il problema è risolto in via definitiva. Circa l'argomento che viene sollevato, secondo il quale, in ogni caso, nella nella posizione della Commissione ci sarebbe comunque un elemento che ricostituisce, per quel che riguarda lo Stretto, una

decida che tipo di futuro intende dare, anche dal punto divista infrastrutturale, al Paese e si metta d'accordo sulle questioni importanti perché il messaggio e l'esempio che dà ai cittadini italiani è veramente devastante.

l'emendamento è stato frutto di una lunga discussione a cui non ci siamo sottratti e che rappresenta comunque, a nostro avviso, una risposta a una scelta che il Governo ha già

Qui si sta discutendo se sopprimere o meno la società Ponte sullo Stretto e lo dico anche a quei colleghi che hanno dei dubbi e che in queste settimane si sono lasciati appassionare dai temi relativi ai costi della politica. Qui siamo davanti a un costo improprio di una struttura che negli ultimi anni, sotto la gestione dell'amministratore delegato Ciucci, che è anche presidente dell'ANAS, è aumentato in modo esponenziale solo per le spese consulenziali. Il ponte

quanto mi riguarda è discutibile, ma la scelta compiuta è di andare allo scioglimento della Società. Ritengo però del tutto sbagliato il comma che riguarda l'istituzione dell'Agenzia, perché penso che siano sufficienti i poteri ordinari dei Ministeri

il mio voto contrario a tutto l'emendamento.

procederò all'organizzazione dei tempi per poter arrivare all'approvazione del decreto nei termini stabiliti.

Le varie legislature hanno visto in tante occasioni il passaggio di colleghi al

l'urgenza della decisione al ministro Bianchi. Presidente, quello che è successo pochi minuti fa credo imponga una riflessione al ministro Bianchi e al Governo. Il Governo è stato battuto su un indirizzo specifico, sul no al ponte sullo Stretto di Messina e sulla cancellazione della società Stretto di Messina.

degli ecologisti e degli ambientalisti. Credo che non possa passare con sufficienza quanto è successo pochi minuti fa in Senato. Il Governo è stato battuto su un problema fondamentale, ossia lo Stretto di Messina e il suo no, che non è stato condiviso dall'Aula. Senatore Strano, da quello che mi risulta - ma potrei sbagliare - il Governo ha vinto e la maggioranza è stata battuta, perché mi risultava che il Governo

Vi sono stati abusi nell'utilizzo di questi strumenti delicati ed estremamente rischiosi. Abbiamo chiesto una verifica, oltre all'istituzione di una commissione di indagine, per capire compiutamente il fenomeno che accresce lo *stock* del debito degli enti locali. poi un debito sommerso, che il ministro Padoa-Schioppa minimizza, anche se non è dato sapere quanto è stato stipulato da banche estere, tramite filiali e filiazioni, per i non residenti in Italia.

Riteniamo che non debbano essere fatti regali alle banche, soprattutto con l'elevazione ad un euro delle commissioni bancarie. intervengo per sottolineare che questa ormai è una legislatura surrealista, perché non si è mai verificato, nella storia di questo Parlamento,

che credo di avere qualche minuto di tempo per rispondere alla proposta del relatore, sul tema sollevato da un emendamento presentato in Commissione bilancio e da ben due interrogazioni parlamentari,

Mi pare che l'emendamento che il relatore suggerisce sia in realtà quello che questo Governo propone, nel tentativo estremo di continuare a coprire il grande scandalo dei derivati che in questo Paese sta assumendo proporzioni assai preoccupanti. Se persino l'ex presidente della CONSOB Rossi ha dichiarato su «Milano Finanza» di due giorni fa

dato la parola.

Presidente, di questo tema abbiamo già discusso in Commissione, su un precedente testo presentato dalla senatrice Bonfrisco, poi riformulato con contenuti molto più impegnativi, nel testo oggi al nostro esame. Avevamo convenuto in Commissione di ricercare un'intesa su questa materia, che ha occupato l'opinione pubblica, il sistema degli enti territoriali e quello creditizio, nonché l'attenzione del Governo. Ritengo che il testo della senatrice Bonfrisco sia eccessivamente

su questi prodotti finanziari (o di autorizzazione o di evidenziazione dei profili di rischiosità e, quindi, di assunzione di responsabilità di chi è chiamato a stipularli). Per queste ragioni, inviterei sia la senatrice Bonfrisco sia il relatore a ritirare questi emendamenti e a convenire di svolgere la discussione sul testo presentato in finanziaria, approfittando di questi giorni per pervenire ad una formulazione condivisa. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il Gruppo di AN ritiene del tutto insoddisfacente la riformulazione proposta dal relatore. Può darsi che, come dice il collega Legnini, ci siano degli elementi, più che invasivi, di dettaglio nell'emendamento 11.0.550 della senatrice Bonfrisco, ma esso è certamente un tentativo di affrontare questo problema. La Commissione ha perso un'occasione per fare questo lavoro che oggi ci propone di fare in finanziaria il collega Legnini.

11.0.1. Vede, Presidente, rispetto alla vicenda che colpisce le famiglie avevamo anche proposto di utilizzare la norma Bersani relativa alla portabilità dei mutui, cosa che non è stata fatta da questo Governo e da questa maggioranza.

la discussione e l'approvazione di una norma più stringente in sede di finanziaria, così come è stato richiesto dal relatore affinché in quella sede possa essere approvata una norma più puntuale.

diventasse una proposta a disposizione dell'Assemblea. Non sono mai d'accordo a rinviare a domani quello che potremmo e dovremmo fare oggi. Il problema degli *swap* e dei derivati è grandissimo grandissimo e investe, al di là di quello che possiamo immaginare, tutte le amministrazioni locali, con amministratori che, a volte per sprovvedutezza o perché sono in qualche modo degli speculatori, spostano il debito dell'amministrazione sugli anni futuri, incidendo così sulla vita futura delle comunità locali. È un problema serissimo che speravo venisse affrontato già in questa sede. Sono d'accordo, quindi, con lo spirito dell'emendamento che la collega Bonfrisco ha proposto all'Aula e mi permetto, signor Presidente, di

perché il problema è più grave e più urgente di quello che si crede. Questa era la sede in cui potevamo e dovevamo trovare un modo per uscire da una situazione di non governo dei fenomeni derivati:

notare che la vera differenza tra la formulazione della senatrice Bonfrisco e quella proposta dal relatore consiste nel fatto la senatrice Bonfrisco definisce obblighi di informazione a carico degli intermediari finanziari che sono previsti adesso dalla direttiva MIFID, finalmente recepita, e che quindi sono ampiamente ricompresi nella riformulazione del testo del relatore laddove si dice che i prospetti saranno redatti a cura di Banca d'Italia e di CONSOB in relazione, naturalmente, alla direttiva MIFID nuova, che fornisce obblighi di informazione e di tutela degli interessi del risparmiatore assolutamente solidi. Quindi, secondo me, se invece di affrontare la questione con tanta animosità si entrasse un momento nel merito si vedrebbe che le differenze tra le due soluzioni sono limitate. Siccome la direttiva MIFID contiene un esplicito divieto di introdurre per gli intermediari obblighi non previsti dalla direttiva stessa, ma cerca di fare in modo che tutti gli intermediari abbiano gli stessi obblighi di conoscenza, la soluzione proposta dal relatore in termini di riformulazione altro non è che l'emendamento della senatrice Bonfrisco, reso compatibile con la direttiva MIFID. Secondo me si potrebbe votare la riformulazione del relatore. la riformulazione del relatore. Se non si fa, perdiamo un'occasione, lo faremo in finanziaria. Tuttavia sarei tranquillo nel considerare i problemi risolti attraverso la riformulazione. Sono convinto che nel merito anche con la senatrice Bonfrisco si potrebbe trovare l'accordo. PRESIDENTE. Ha chiesto

per quanto riguarda la gestione e la programmazione in ambito scolastico. L'emendamento 12.5 vuole evidenziare in particolare il fallimento della politica di contenimento dei costi e della riduzione del personale,

una modifica testuale di una legge, quindi bisogna fare chiarezza, mettere un punto fermo qual è, appunto, quello indicato nell'emendamento 13.1.

Chi è senza peccato scagli la prima pietra, da una parte e dall'altra. Passiamo

su questo emendamento che, tra l'altro, ha una sua genesi strana e un risultato particolare. Lo stesso provvedimento, almeno nella *ratio*, è già previsto nella finanziaria dello con tempi che non sono probabilmente quelli che tutti noi auspicavamo, ma il processo di razionalizzazione delle scuole della pubblica amministrazione è in corso. Ora, il Parlamento, non contento evidentemente dell'azione iniziata sulla base della legge finanziaria dello scorso anno, sanziona in maniera perentoria il Governo, imponendogli, nell'amplificare peraltro alle scuole speciali come l'Istituto diplomatico e la Scuola per prefetti, una data che è per lo meno fuori dalle consuetudini: si provvede cioè a chiudere queste scuole nel momento in cui questa legge verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Io credo che ci sia uno stato d'animo o un sentimento nei confronti di questa vicenda che dovrebbe essere riportato alla razionalità. Non è questione di parte, opposizione o maggioranza, è un appello che faccio anche al Governo, al quale devo dire, peraltro, che capisco che il non sia interessato alle scuole, però forse anche ascoltare il parere di componenti di altri Ministeri l'avrebbe portato a non dare un parere favorevole a questo oltretutto, non solo questo vuol dire smantellare un patrimonio di scuole di formazione ministeriali ma anche, molto probabilmente, impedire che si possa attuare quella razionalizzazione che la legge finanziaria dello scorso anno prevedeva. Quindi, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale, invito anche gli altri Gruppi a ragionare; ripeto, non è una questione di parte, è una questione che riguarda le strutture della pubblica amministrazione: siamo per la qualità dei funzionari e stiamo provvedendo ad eliminare le scuole di formazione dei quadri della pubblica amministrazione. Signor Presidente, io vorrei esprimere il mio consenso alla posizione della Commissione e il mio apprezzamento per il parere del relatore e del Governo. Mi consenta una brevissima premessa: noi abbiamo nel nostro sistema una molteplicità di scuole, scuolette e scuolettine, anche in specie ministeriali, per la formazione del personale pubblico.

di questa iniziativa parlamentare è di riprendere una strada che si era

il quale ha inteso banalizzare una tradizione assai consolidata nella formazione dell'alta burocrazia del nostro Paese, sottacendo il tentativo di smantellamento delle scuole dei singoli Ministeri (che fiori all'occhiello della nostra istruzione anche in campo europeo ed hanno prodotto la possibilità di raccordi e di istruzione, soprattutto negli ultimi anni, per i Paesi che hanno contraddistinto l'allargamento dell'Unione Europea e che sono venuti alle nostre fonti, alla nostra tradizione del diritto) e anche dell'alta burocrazia, la cui valenza ho avuto modo di toccare direttamente con mano. La La banalizzazione del senatore Villone ha trascurato di dire che l'accentramento in un'unica Agenzia rappresenta ancora una volta un segnale di questo Governo di voler demolire l'esistente per gestirlo secondo le direttive di qualcuno, di qualche singolo esponente dell'Esecutivo.

se tornare indietro rispetto ad un orientamento già assunto con la precedente finanziaria e che prevede la razionalizzazione del sistema formativo, come capita in molti Paesi europei (l'esempio francese su tutti). Qui c'è una questione specifica che riguarda che cosa succede nella fase in cui non è ancora entrato in vigore il regolamento. Sotto questo profilo, avevo presentato un disegno di legge, su cui la 1a Commissione permanente si era espressa in modo largamente favorevole, il quale tendeva appunto a far sì che la scuola resti in vita sino al momento in cui viene approvato il regolamento. Quindi, possiamo esaminare la questione solo sotto questo profilo, non caricandola di significati politici che non ha. L'emendamento della Commissione può essere condiviso o meno, ma non si tratta di rimettere in discussione un orientamento già maturato in Parlamento.

circolare in tale direzione. Non comprendo allora questa accelerazione: si tratta di favorire qualcuno che aspetta di diventare il grande direttore generale di un'immensa scuola di formazione?

Signor Presidente, siamo di fronte all'ennesimo tentativo da parte del Governo e della maggioranza, almeno di una buona parte di essa, di sopprimere alcune istituzioni importanti del nostro Paese e concentrare in un'unica soluzione di potere, questa fantomatica Agenzia,

una storia che vuole chiudere la Scuola superiore della pubblica amministrazione, che vuole sopprimere l'Istituto diplomatico ed altri enti importanti.

che denunceremo come atto di vandalismo politico che si sta perpetrando nei confronti di istituzioni del nostro Paese.

il Governo sta lavorando alla formulazione del regolamento che dovrebbe dare attuazione alla norma contenuta nella finanziaria dell'anno scorso. Rinnovo tale appello; in caso negativo il

desidero sottolineare che il Gruppo UDC voterà contro l'emendamento della Commissione, soprattutto sapendo che il Governo non ne fa una questione di maggioranza di Governo: è una questione politica di Aula,

già in Commissione abbiamo avuto modo di puntualizzare la nostra posizione su questo emendamento, che è frutto di una proposta della maggioranza approvata a maggioranza dalla Commissione e che riguarda

che siamo già al secondo anno e che sono fortemente avanzati i lavori per creare un grandissimo centro di ricerca biotecnologica a Palermo.

se ci sono cose da segnalare in tutte le direzioni la Presidenza ha intenzione di far rispettare il voto nominale.

Mi appello, però, al senso istituzionale del ministro Mastella per invitarlo, visto che risulta votante mentre in effetti non era in Aula, a riconoscere questo dato. Invito la Presidenza, alla luce dell'eventuale chiarimento del ministro Mastella, a ripetere la votazione. Signor Presidente, può succedere qualche incidente di percorso, ma quando viene fatto votare un componente del Governo che non è in Aula, credo che ne pianga

esponenti del Governo votano mentre non sono in Aula, venga corretto con un chiarimento ed una ripetizione della votazione. sa, senatore Schifani, sa che in questo periodo sono costretto a difendermi da diverse schifezze. Debbo dire, però, con molta obiettività,

Presidente, non ho alcuna difficoltà a riconoscere che lei guida i lavori di quest'Aula con molto garbo e con molta attenzione. Però in questo momento siamo in una situazione molto delicata, perché in Aula su ciascun emendamento si perde o si vince per un voto. voto. Com'è ovvio, la giustificazione del ministro Mastella non ha alcun senso; se la accettassimo per modificare la scelta di voto, significherebbe che ciascuno di noi si può alzare e spiegare perché c'era o perché non c'era. Resta però un fatto: nella votazione precedente,

che in un momento come questo è importante più per la maggioranza esserci, per non essere battuta, che per l'opposizione tentare di fare il pianista. avviso, qualunque ritardo che lei agevola nel ritenere chiuso il voto, di fatto, altera quello che in quel momento può essere il risultato finale, come, ad esempio, è avvenuto poco fa. fa. Pertanto, la voglio pregare da questo punto di vista di avvertire preliminarmente, se lei lo ritiene, tutti i parlamentari ad essere attenti al voto che si sta per esprimere

sostanzialmente per quel voto che il ministro Mastella ha testé affermato di avere espresso, per poi allontanarsi e rientrare in Aula una volta...

Il ministro Mastella è rientrato dopo che era stata dichiarata chiusa la votazione. In assenza di quel voto, Presidente, quell'emendamento non sarebbe passato e per l'ennesima volta oggi la maggioranza sarebbe andata sotto. Ma non è questo il problema, signor Presidente. Volevo rappresentarle che ieri, nel corso di una votazione, ho espresso il voto, sono uscito e, in ragione di un'evidente e ridotta mobilità rispetto al ministro Mastella, non ho fatto in tempo a riposizionarmi per confermare l'espressione del voto. In ragione di tutto questo, in una situazione analoga la Presidenza la Presidenza - immagino su invito del solerte amico e segretario di Presidenza, senatore Ladu - ha imposto al senatore Mauro di estrarre la mia scheda.

Faccio altresì presente di avere già sollevato in passato questo problema quando, in riferimento ad un emendamento bocciato dall'Aula, il presidente Marini ha inteso far ripetere il voto e il giorno dopo il vice presidente Angius, che era Presidente, non ha adottato uguale provvedimento in una situazione analoga. Tutti quanti noi sappiamo qual è la situazione

di salvaguardare l'istituzione che ella in questo momento rappresenta. Consenta a me, come senatore della Repubblica, di manifestare il mio più profondo rammarico per questa disparità di trattamento che ha caratterizzato le decisioni della Presidenza e che per la seconda volta, senza che lei, Presidente, ne abbia colpa alcuna, ha oggettivamente favorito la maggioranza maggioranza riscaldando quel brodino di cui ha avuto modo di parlare il Presidente della Camera in una sua intervista.

credo abbia aperto le porte (ed è quello che noi faremo) ad una possibilità - direi un *vulnus* proprio nel comportamento - nel momento del voto da parte dei senatori del seguente tipo: in sostanza, posso votare,

nel momento in cui, avendo votato regolarmente prima della nostra uscita dall'Aula, rappresenteranno un voto in un senso o nell'altro rispetto a quanto siamo stati chiamati a votare. Credo sia molto grave che che lei non abbia fatto togliere, nonostante l'appello del presidente Castelli, la scheda del ministro Mastella, e altrettanto molto

mi aggiungo alle tante vestali della legalità che sono apparse in quest'Aula, tutte vergini che vedono violata la loro legalità. Mi permetto, da una postazione privilegiata - sono quello che sta, come tanti, più in alto di tutti di rammentare che due senatori del centro-destra sono entrati in Aula dopo la votazione.

La scoperta che si fa quotidianamente, insieme a tutti gli organi di informazione, del fatto che al Senato la maggioranza, ove ci sia, ha un voto o due in più dell'opposizione, mi sembra la scoperta della cosiddetta acqua calda e ciò accade tutti i giorni.

Non si può restare in piedi mentre si vota perché ciò significa inesorabilmente occultare un voto illegale espresso dietro. Questo succede nel centro-sinistra e nel centro-destra. Se il Presidente di turno non decide che tutti devono essere seduti prima di proclamare il voto e non fa il controllo relativo, non se ne viene a capo in nessun modo. Una volta avrà ragione l'uno,

nell'esame di questo provvedimento, se non si chiarisce questo punto, dati i risicati limiti che ci sono fra la maggioranza e l'opposizione. Pertanto, le chiedo formalmente, Presidente, di riunire immediatamente la Giunta per il Regolamento, affinché si pronunci sull'argomento. A quel punto, potremo proseguire i nostri lavori. Signor Presidente, durante la crisi dell'Impero romano d'Oriente, i saggi a Bisanzio discettavano sul sesso degli angeli.

Questo è l'unico modo con cui oggi possiamo tranquillamente

torna in Aula eppure quel voto è valido. Se lei fa passare questo precedente, si annullerà ogni controllo sui cosiddetti pianisti, perché ciascuno di noi potrà votare per gli altri e uscire dall'Aula. Così lei non potrà mai controllare come si vota.

la scheda del ministro Mastella. Lei non ha voluto guardare dove le indicava il presidente Castelli e questo è molto grave da parte di chi presiede l'Aula.

gli credo. Egli dichiara di aver votato e di essersi poi allontanato, non ho motivo per non credere alle parole del Ministro, persona che tra l'altro stimo. Comunque, il ministro Mastella, con la sua onestà, ha aperto un tema,

alla *buvette*, considerando che il proprio voto è validamente dato? Questo è il tema che poniamo. Signor Presidente, riconosciamo che in tutte le votazioni sono state sottratte delle schede dove si manifestava un'espressione di voto perché non si individuava all'interno dell'emiciclo la presenza del senatore. Quante schede sono state sequestrate proprio perché si è riscontrata l'assenza materiale del parlamentare al quale corrispondeva la scheda? altro aspetto, vorrei rifarmi all'intervento accorato e responsabile del presidente Morando. Il presidente Morando ha posto il tema dell'assegnazione dei posti. Ce ne occuperemo, però, per cortesia, di cosa stiamo parlando? Abbiamo preso atto che oggi in questa Aula la maggioranza è andata sotto, non per episodi banali di pianismo, non per episodi di voti espressi da senatori che non erano in Aula, ma soltanto perché pezzi della maggioranza hanno votato significativamente con l'opposizione.

di ambulantismo senatoriale, chi c'è vota e chi non c'è vota lo stesso. Il tema che oggi sta esplodendo in questa Aula in tutta la sua evidenza è il seguente: non c'è più una maggioranza politica per il semplice motivo che su temi significativi vi siete dilaniati, vi siete divisi e vi siete spaccati. sono state fatte diverse valutazioni. Devo dire francamente, in uno spirito che credo possiate capire, che mi hanno colpito non già le valutazioni su un possibile errore della Presidenza, che ovviamente è sempre

la votazione in tempi un po' differiti perché i senatori segretari, facendo il loro lavoro, quindi non è loro responsabilità, mi avevano segnalato dei casi che dovevano essere valutati. Da questo punto di vista, mi che la questione sia chiara e non ho intenzione di accettare alcuna valutazione di disparità di trattamento, perché anch'io ieri ho assistito alla vicenda che ha riguardato il senatore Palma.

possa avvenire solo in presenza del senatore o della senatrice in Aula. Questo non è un luogo di passaggio dove uno vota e poi va a fare telefonate, va alla *buvette* o anche a svolgere altri compiti. Per questi motivi,

ripetere, con un gesto importante e anche un po' irrituale, che il voto si esprime solo in presenza del senatore e della senatrice, annullo il voto precedente e dichiaro nuovamente aperta la votazione.

Presidente, lei ricorderà che il risultato della votazione è stato 157 e 156 ed in quel momento, come tutti hanno riconosciuto,

ma la sua posizione è stata eccessivamente accomodante. Come vede, poi, il risultato è stato quello che è stato. Si è disquisito troppo sulla questione del voto, mentre la realtà sostanziale è un'altra:

di provvedimento e di deliberazione avessimo assunto non avrebbe avuto alcun significato effettivo. Con questo emendamento, noi chiediamo semplicemente che il lavoro dell'ARAN sia svolto su risorse effettivamente stanziate in finanziaria e, qualora vi siano accordi aggiuntivi, che questi avvengano nel momento in cui le risorse sono state reperite.

sull'emendamento 15.0.2 che, in Commissione, è stato bocciato perché mancante di copertura così non è perché questa proposta emendativa è relativa all'assunzione di dirigenti già assunti in seguito a provvedimenti dei giudici del lavoro e risultati idonei al concorso per dirigenti del Ministero della giustizia, bandito con un provvedimento del Direttore generale del Ministero della giustizia il 13 giugno 1997. Peraltro, l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i dirigenti di cui in premessa già prestano servizio presso gli uffici giudiziari in forza di provvedimenti cautelari; anzi, porta un risparmio di spese da parte del Ministero della giustizia, in quanto l'inquadramento in via definitiva farebbe venir meno il contenzioso, con evidente risparmio per il bilancio dello Stato.

aiutare la soluzione di un problema che ormai nella pubblica amministrazione costituisce un fondamentale principio di diritto. Vorrei sottolineare che vi sono circa 7.500 dipendenti pubblici a tempo indeterminato, assunti con regolare concorso, che sono comandati nella pubblica amministrazione e ricoprono ruoli ormai fondamentali, strutturali

a non essere inquadrate, ad essere soltanto comandate; quindi, l'ordine del giorno - non abbiamo voluto presentare un emendamento per non caratterizzare questo intervento questo intervento - vuole impegnare il Governo a studiare una soluzione, che noi immaginiamo sia quella di regolamentare e regolarizzare queste 7.500 persone,

mi atterrei agli orientamenti non contestati del mio predecessore; quindi, vi prego di svolgere interventi molto brevi in modo da poter raggiungere un risultato apprezzabile nella votazione del provvedimento.

delle tre carte e dice che bisogna restituire potere al Parlamento perché il Parlamento non sarebbe nelle condizioni di esercitare il potere di indirizzo e di decisione. In questo caso si tratta, appunto, delle procedure relative ai contratti della pubblica amministrazione. Sappiamo tutti che, di solito, la procedura è questa: il Governo inserisce in finanziaria

potrebbe benissimo essere ritirato, perché non porta modifiche sostanziali alle procedure che di solito vengono adottate. In ogni caso, se non viene ritirato, il parere è contrario.

Presidente, intervengo su un emendamento che mi ha un po' incuriosito e spero non incuriosisca tutti i cronisti che si occupano di antipolitica.

che propone la stabilizzazione di certi rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, ma di essere incline a suggerire al Governo di accogliere quest'ordine del giorno come raccomandazione. Lei sa, e non devo spiegarla all'Aula, qual è la differenza.

il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 17 ottobre-14 novembre, così come deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo il 17 ottobre. È stato comunicato che per quanto riguarda il provvedimento in questione i tempi sono contingentati. Ho qui

Presidente, in questa votazione c'è stato addirittura un collega dell'opposizione che ha sbagliato e per Quindi noi saremmo dovuti essere 158. Tutti i colleghi dichiarano di avere votato, Presidente. *(Proteste Presidente, aspetto il tabulato dal quale risulterà che due colleghi della maggioranza non hanno votato. Si alzeranno i due colleghi e diranno che non è vero. Loro hanno partecipato alla votazione, perché si sa che i numeri sono questi e

era al telefono e non ha fatto in tempo a votare. Si è poi meravigliato del fatto che una volta chiusa la votazione non abbia potuto votare. Ricordo al collega che anche quando si guida con il telefonino in macchina si perdono

Ora siamo persino arrivati a sostenere che qui qualcuno trucca il voto. Mi pare un po' eccessivo fare questa considerazione. prende la parola e chiede di verificare per perdere tempo, perché è evidente a tutti che la sua maggioranza è in un momento di crisi. È ovvio che «momento di crisi» è un eufemismo, perché questo momento dura da un anno e mezzo. mezzo. Questa è la verità, e allora vorrei pregare la Presidenza di non prestarsi a questo ostruzionismo surrettizio. Sicuramente dobbiamo dare atto dell'abilità del collega Boccia.

intervengo soltanto per informare. Capisco l'animosità di tutti qui accanitamente schierati, tra cui il sottoscritto, per il voto in più o il voto in meno. Vorrei solo far notare che tutti gli emendamenti della Commissione all'articolo 16, compresi quelli che stiamo per votare, sono emendamenti sì approvati dalla Commissione ma su testi proposti dall'opposizione. Quindi, capisco tutto, ma attribuire un significato politico al fatto che un emendamento dell'opposizione accolto dalla Commissione non venga approvato dall'Aula è,

la maggioranza, che ha già votato a favore all'unanimità in Commissione, confermerà il suo voto. Se nel frattempo l'opposizione ha cambiato opinione su quegli emendamenti e non li sostiene più, pazienza non passeranno, ma non succede niente di politicamente rilevante.

non nascondo la mia grande ammirazione per il senatore Morando. Non la nascondo, però delle volte l'abilità è superiore agli effetti che intende produrre. Lui è venuto a dire che se noi votiamo e la maggioranza no, la maggioranza avrebbe ugualmente il diritto di ritenere di

per un effetto traslativo. Capisco l'abilità però anche il funambulismo ha i suoi limiti.

Presidente, non avrei chiesto di parlare se non fosse intervenuto il collega Morando prima. Non è assolutamente vero che in Commissione sono stati approvati normalmente degli emendamenti dell'opposizione. Il caso politico sia dello Stretto di Messina, sia della scuola superiore c'è ed è clamoroso. Il senatore Morando non dica cose non vere. Qualche emendamento della Commissione è dell'opposizione, ma questo rappresenta un caso politico

dichiaro aperta la votazione. Mettetevi seduti perché la regola vale per tutte le sedute non per una sola.

Non mi soffermo sull'importanza di questa vicenda più volte richiamata in quest'Aula. Con l'emendamento 18.2 pongo il problema di una salvaguardia rispetto a quanto sta accadendo con l'ICI.

chiedere fino a cinque anni di arretrati. Questa misura è particolarmente odiosa perché il beneficio che questo Governo prevede in favore dell'ICI viene assolutamente vanificato con una richiesta di tale portata.

in maniera significativa la grave crisi di redditività che sta in questo momento interessando le imprese del settore della pesca del nostro Paese. A lei e ai colleghi sarà noto che, dato l'atteggiamento remissivo e rinunciatario del Governo Prodi, a Bruxelles è stata approvata una riforma del settore della pesca mediterranea che introduce delle innovazioni fortemente penalizzanti per un settore in crisi di redditività. Aggiungo che l'aumento del prezzo del petrolio e dunque del gasolio

delle norme relative alla trasmissione telematica dei dati, gli intermediari finanziari hanno trovato difficoltà per causa a loro non imputabile. Con questo emendamento, che non costa nulla, si dà la possibilità a costoro, che sono grandi ausiliari, e che da soli hanno consentito la costruzione dell'anagrafe tributaria, di ripetere senza sanzioni l'adempimento.

ripropone la rottamazione, che era stata introdotta con la scorsa finanziaria.

sopprimere gli articoli 18 e 41. Ricordo che l'articolo 18 è molto importante, poiché interviene sugli adempimenti conseguenti agli impegni internazionali. Vi sono alcuni interventi significativi per quanto riguarda gli accordi di pace ed altri interventi molto importanti che riguardano la partecipazione italiana al sostegno ai Paesi in via di sviluppo. Con riferimento agli accordi di pace,

18.8 è importante e riprende in generale il tema degli interventi a sostegno

l'inserimento nel decreto di una norma che era stata stralciata dalla finanziaria, inerente ad un intervento a favore delle vittime del mare. Su questo intervento c'è un parere uniforme da parte dei membri della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione. Credo si tratti di un intervento significativo,

Mi dispiace che anche rappresentanti del Gruppo dei Verdi si muovano in senso contrario a quello che dovrebbe invece essere un obbiettivo comune. Si pone, dunque, la necessità di far crescere e di determinare uno sviluppo forte e in modo competitivo.

di 500 milioni di euro per interventi per la pace e lo sviluppo. Il Governo italiano si impegna, tra l'altro, a sostenere la *Peace Facility*, cioè una struttura di finanziamento per la gestione di operazioni di pace in Africa, e quindi di sviluppo delle capacità endogene dei Paesi africani di intervenire con propri contingenti militari di pace. Si tratta di un aspetto estremamente importante: pensiamo, ad esempio, al caso del Darfur, che richiede un impegno forte da parte dei Paesi di quel continente per portare pace in quella zona. zona. Vorrei richiamare poi anche il contributo di 130 milioni di euro per la costituzione di un Fondo globale contro la malaria e l'AIDS, che si aggiungono ai 260 già stanziati dal Governo, e che dovrebbero andare ad anticipare la rata per il 2008, tenendo quindi finalmente fede ad un impegno che da troppi anni era rimasto disatteso.

del Gruppo dell'Ulivo. Non ho alcuna intenzione di far perdere tempo all'Aula, ma voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sulla portata particolarissima di questo emendamento.

Diciamo la verità, non abbiamo sempre onorato con precisione questi impegni, né quando abbiamo governato noi, con i Governi di centro‑sinistra, né nella fase del Governo di centro‑destra.

di 100 milioni di euro per l'ONU, per le forze di pace e per la Corte penale internazionale. Richiamo solo questi due esempi per indicare la portata straordinaria di questi impegni, che non sono della maggioranza contro l'opposizione, o viceversa.

per il nostro Paese è moralmente inaccettabile sopprimere l'articolo 18, che

che reca una dotazione di 150 milioni destinati all'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa

aiutare l'industria e favorire un minore inquinamento possa essere apprezzabile,

vorrei rivolgermi con il cuore in mano al collega Eufemi perché ritiri questo suo emendamento, che in sé può essere naturalmente discusso come una proposta interessante, ma non in questa sede e non in alternativa a questo finanziamento agli adempimenti conseguenti ad impegni internazionali. Credo non sfugga a nessun collega, tanto meno ai colleghi dell'UDC che su questo hanno una storia anche di attenzione alla solidarietà internazionale, quanto sia significativo ed importante. Vorrei anche rendere noto all'Aula che su questo punto c'è stato un consenso unitario all'interno della Commissione affari esteri, che ha espresso un parere favorevole veramente con il plauso e il consenso di tutti, Senatore Tonini, vorrei pregare non lei, che sta parlando regolarmente,

Come Gruppo di Alleanza Nazionale condividiamo gli obiettivi che si pongono in questi emendamenti. Non condividiamo, però, che la copertura venga trovata attraverso la soppressione dell'articolo 18, perché questo mette in difficoltà gli impegni internazionali del Paese, e non è un problema di maggioranza o opposizione. Pertanto, vorrei chiedere al collega Eufemi se accedesse ad una riformulazione sulla copertura, onde evitare che questi emendamenti vadano a togliere le risorse all'articolo 18 per gli impegni internazionali dell'Italia. In caso contrario saremmo costretti a votare contro, non per il merito dell'emendamento, ma per la formula scelta per la copertura. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti. Non ho nessun problema a modificare la copertura in questo senso. Era una copertura esclusivamente tecnica, tant'è vero che anche la norma

sufficiente ricorrere all'articolo 41, che è quello della società di scopo immobiliare, per coprire abbondantemente l'emendamento, perché il costo è di 100 milioni di euro e lì ce ne sono 150. escludiamo pure la questione delle missioni internazionali, sulle quali certamente non volevamo intervenire. Si trattava soltanto di un problema di copertura tecnica

Non è vero che l'articolo 18 intervenga su spese obbligatorie: ci sono molte spese che incidono su ulteriori finanziamenti, sulla costituzione di nuovi capitoli, sui contributi volontari. Qui non si tratta,

*(Aut)*. Signor Presidente, vorrei chiarire in tutta serenità un aspetto politico che non può essere archiviato senza averlo opportunamente chiarito.

Nella discussione del testo avevo pensato di mettere una "o" al posto della "e" per introdurre un elemento di maggiore chiarezza. Nel merito ho però ricevuto le rassicurazioni da parte del Governo, del presidente della Commissione bilancio e del relatore sul fatto che il testo così come era scritto andava bene, in quanto riprendeva la dizione originale della legge in vigore. Tale legge, la n. 250 del 1990, è stata sempre applicata nel senso da me esposto, vale a dire che le radio fanno informazione nella lingua della minoranza linguistica che rispettivamente rappresentano.

Ritengo che sia un fatto grave e offensivo della nostra Carta che una prerogativa prevista nei princìpi basilari sia delegata ad una istanza, come è stato detto, localistica e campanilistica.

C'è stata una decisione sconcertante, cioè una sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, previa emissione di una ordinanza in materia di documenti coperti da segreto di Stato.

all'apposizione del segreto di Stato in questa vicenda e in quella del sequestro di Abu Omar. Questa vicenda, e quindi la sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sull'omicidio Calipari, non è soltanto una rinuncia alla giurisdizione, ma una grave rinuncia alla sovranità nazionale. Pensavo che certi tempi e certe soggezioni, anche giuridiche, fossero soltanto del passato: evidentemente non è così. Con questa decisione della Corte di assise di Roma si è rinunciato alla ricerca della verità. Confidiamo che gli gli organi dello Stato, e in particolare il pubblico ministero, formalizzino un'istanza di ricorso in Cassazione per eliminare una vera e propria ingiustizia e una rinuncia alla verità.

dell'Aula e della Presidenza su una vicenda molto grave. È in corso di svolgimento, davanti alla prefettura di Napoli, una manifestazione di centinaia di cittadini, con la partecipazione di parroci, mamme, donne e bambini dell'area giuglianese, per protestare contro la decisione del commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania di prorogare l'apertura e il funzionamento del sito di stoccaggio di Taverna del Re, nel Comune di Giugliano. Signor Presidente, ho presentato un'interrogazione urgente (la esattamente a giugno, in occasione dell'approvazione del decreto-legge sull'emergenza rifiuti in Campania, aveva votato un ordine del giorno con il quale si stabiliva in maniera tassativa che il termine finale per l'attività di stoccaggio nel sito Taverna del Re nel Comune di Giugliano fosse il 31 ottobre